Onorevoli colleghi, il 23 maggio 1992,

dove fare soltanto il proprio dovere assume una connotazione di rischio. Giovanni Falcone era un magistrato di altissime doti e di eccezionale intuito investigativo. Egli aveva prima di tanti altri compreso che soltanto il contrasto efficace e concreto alla mafia avrebbe potuto contribuire alla rinascita complessiva della sua terra. Per questo, fin dall'inizio della sua esperienza di magistrato a Trapani e successivamente a Palermo, aveva dedicato interamente la sua vita professionale a comprendere il fenomeno mafioso, nella piena consapevolezza che soltanto una profonda conoscenza dei meccanismi di questa organizzazione criminale avrebbe potuto contribuire a scardinarla dall'interno. E da giudice istruttore aveva avuto la grande intuizione che soltanto lavorando in sinergia e coordinamento con gli altri giudici che si occupavano di indagini sulla mafia si sarebbe potuto realizzare quel modello veramente efficace per contrastare un'organizzazione verticistica, gerarchica, unitaria, che operava nelle scelte decisive con coesione e comunione di intenti. Così era nato il *pool* antimafia, scelta rivelatasi da subito vincente, allorché il primo grande collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta, aveva chiesto di parlare proprio con Giovanni Falcone ed aveva disvelato i meccanismi interni dell'organizzazione Cosa nostra. Da allora erano iniziati i grandi processi: il maxiprocesso del 1986, con centinaia di imputati alla sbarra, aveva segnato il primo grande momento di contrasto a questa organizzazione criminale. Aveva significato il primo grande riconoscimento dell'esistenza del reato di associazione criminale di stampo mafioso, ingenerando tra i mafiosi la grande preoccupazione, rivelatasi fondata, che quello era un momento di non ritorno. E poi le condanne severe, inflitte grazie alla serietà ed alla capacità investigativa di questo grande giudice, avevano fatto ulteriormente comprendere ai mafiosi che da quel momento sarebbe stato sempre più difficile poter operare liberamente nell'impunità. Falcone non aveva mai smesso di credere nella sua intuizione, neppure quando aveva ricevuto da parte di tanti, che avrebbero invece dovuto riconoscerne e proteggerne il valore, insinuazioni e pesanti critiche che tanto lo avevano addolorato. Neppure quando aveva scelto di divenire Direttore generale degli Affari penali a Roma, decisione, questa, che era stata interpretata come una volontà di abbandono della Sicilia e che invece, nelle sue intenzioni, come non smetteva di dire ai suoi collaboratori più fidati, rappresentava un ulteriore più efficace modo per poter continuare a combattere la mafia. Falcone era stato un grande sostenitore della necessità di concentrare le indagini nelle procure sedi delle corti d'appello; le Direzioni distrettuali antimafia diventarono una realtà grazie alla sua capacità di rappresentare al legislatore le grandi potenzialità che queste strutture avrebbero potuto estrinsecare. Oggi noi traiamo i frutti benefici della sua caparbia intuizione e ogni risultato attuale, che può sembrare scontato, naturale conseguenza delle cose, va, invece, ricondotto al grande progetto dì Falcone. Ecco perché il nostro ringraziamento a questo eroe dello Stato non deve rivolgersi soltanto al passato, ma deve considerare anche i traguardi del presente. Accanto a Giovanni Falcone, un ricordo commosso va a Francesca Morvillo. Chi ha avuto il privilegio di conoscerla, ricorda di questa donna magistrato, sostituto procuratore al tribunale per i minorenni di Palermo, la profonda conoscenza giuridica ed umana del delicato settore dei minori, la sua grande fermezza di carattere, ma al contempo la sua grande umanità. Francesca Morvillo ha operato per anni non soltanto per reprimere i reati, ma soprattutto per cercare con ogni mezzo di recuperare i tanti minori sbandati e per restituirli ad una vita diversa, migliore, lontana da quelle complicità e quei facili guadagni che in Sicilia costituiscono l'anticamera per l'ingresso in Cosa nostra. Un metodo portato avanti con determinazione e fermezza, in silenzio, un grande contributo anche questo alla lotta alla criminalità. Un ricordo non formale di gratitudine va anche ai tre giovani uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita interpretando fino in fondo un ruolo indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo finale. Abbiamo il dovere della memoria, ma anche quello di vigilare, di essere attenti e di contribuire con la nostra attività di senatori a fare in modo che leggi sempre più efficaci e incisive possano fornire agli inquirenti veri ed effettivi strumenti per contrastare il fenomeno mafioso. Mi riferisco, colleghi, alle disposizioni legislative sulle misure di prevenzione patrimoniali e sull'inasprimento del carcere duro che il Senato si appresta ad esaminare. Dopo la strage di Capaci e ancora dopo quella in cui caddero per mano mafiosa Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta, le forze dell'ordine, la magistratura hanno lavorato con grande professionalità e competenza e molto è stato fatto. Certo, non possiamo ancora affermare che la mafia sia un fenomeno non più attuale. II percorso perché questa affermazione diventi una splendida realtà non è ancora ultimato. Oggi dobbiamo contribuire tutti a fare in modo che la strada tracciata da Giovanni Falcone prosegua fino a piegare definitivamente la criminalità organizzata. Tutti significa ciascuno, significa che non vi sono ruoli secondari nella lotta alla mafia. Dal semplice cittadino all'imprenditore, al politico, ciascuno ha questo compito attivo, ogni giorno, in ogni luogo. E' il solo modo efficace di onorare Giovanni Falcone e gli altri martiri, ma è soprattutto il modo più alto di amare i nostri figli e la nostra Patria.

Signor Presidente, mi riconosco pienamente nelle parole che lei ha pronunziato con l'autorità dell'altissima carica che ricopre. Ci ha rappresentato con le sue parole manifestando dei sentimenti autentici che noi condividiamo. La storia giudiziaria del nostro Paese ci ha ormai consegnato il fatto che il 20 febbraio 1992 la commissione provinciale di Cosa nostra, all'indomani dell'esito del maxiprocesso - esito nefasto per Cosa nostra, non tanto per le condanne quanto per l'annullamento delle assoluzioni - deliberava di sferrare l'offensiva stragista nei confronti dello Stato attraverso l'individuazione degli obiettivi da abbattere, attraverso la triplice indicazione consacrata negli atti processuali: uccidere i nemici; uccidere gli ex amici per sovravvenuta inaffidabilità; uccidere i traditori. Il primo di quei nomi era quello di Giovanni Falcone, già condannato a morte negli anni precedenti, quando proprio attraverso il maxiprocesso aveva concretizzato la possibilità di contestare - ed era un fatto raro che non avveniva da anni

dell'attentato - era un nemico pericoloso, un nemico da abbattere, per tre aspetti significativi che Cosa nostra aveva colto: il suo metodo di lavoro; il suo intuito; la sua capacità di organizzare il lavoro di squadra.

direzione, oltre che con il lavoro fatto con il maxiprocesso - che rimane una pietra giudiziaria fondamentale nella ricostruzione di quegli avvenimenti - attraverso l'intuizione della costituzione della DIA come giustamente si ricordava, della procura nazionale antimafia, delle procure distrettuali e della legge sui collaboratori di giustizia, in un momento in cui l'Italia era veramente in ginocchio (tutti ricordiamo lo sgomento che colse il popolo italiano di fronte a ciò che stava avvenendo ed all'incapacità di individuare una risposta): metodo, modello e strumenti che il mondo ci ha invidiato e ci invidia.

era fedele ad una sua profonda convinzione: la mafia, come tutte le cose umane, è destinata a finire. Con questo Giovanni Falcone voleva dire che combattere la mafia significa impegnarsi con costanza, con intelligenza, con dedizione, con esempi e coerenza, senza arretrare un attimo, perché certe cose finiscono se l'uomo vuole che finiscano e noi come politici abbiamo il dovere di farle finire. Ecco perché è giusto ricordare Giovanni Falcone, ma ricordarlo significa ricordare il suo metodo e i suoi strumenti di lavoro, la sua intelligenza, il suo intuito. Rendere attuale il ricordo di Giovanni Falcone significa rendere attuale la lotta alla alla mafia per poterla sconfiggere, perché dipende da noi.

ne ricordiamo oggi le figure esemplari, l'ammirevole abnegazione, il fulgido coraggio nella lotta strenua e generosa contro il flagello della mafia. doverosa: in questo senso, risulta lieve il peso del pur immenso debito che lo Stato, le istituzioni e l'intera comunità civile hanno contratto nei confronti di chi offrì tutto di sé per la salvezza e il riscatto della propria gente. Da 17 anni per quanto riguarda i martiri della strage di Capaci, ma ormai da mezzo secolo, a datare dalla rimpatriata di Cosa nostra, lo Stato italiano ha dichiarato ostilità aperte nei confronti di mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita. Oggi la mafia siciliana, avendo subito colpi durissimi, cede terreno, che tuttavia viene presto riconquistato alle attività criminose dalle organizzazioni sorelle, *in primis* la 'ndrangheta calabrese. L'immigrazione incontrollata nel nostro Paese, caldeggiata non per virtuoso altruismo cristiano, ma per vizioso masochismo, ha poi consentito la penetrazione in forze di terribili mafie straniere, attualmente soprattutto impegnate a intessere quelle reti logistiche criminali che preludono a sviluppi preoccupanti. La ricorrenza della strage di Capaci è una pietra che si abbatte sulla nostra memoria e sulla nostra coscienza: il doveroso omaggio a Giovanni Falcone non si può esaurire in un rituale, sia pur sentito, celebrativo di un autentico eroe del nostro tempo. C'è la sua lezione, ancora oggi attualissima, che deve essere declinata ai nostri giorni, laddove i segni dell'attività mafiosa sono sempre più visibili, anche in territori lontani dalla culla naturale, e in forme diverse e più raffinate avvelenano e ipotecano pesantemente attività economiche e commerciali del Nord e di ogni parte d'Italia. In questo senso, mi sento di ringraziare il Parlamento, il Governo ed il ministro Maroni, che tiene alta la guardia e provvede a monitorare la progressiva espansione della nuova mafia e della 'ndrangheta, che vanno intrecciandosi dove c'è profumo di affari. Ricordando Falcone, cogliamo una stagione dolorosissima della storia del nostro Paese, quella calda estate che tolse al Paese due formidabili e indomiti servitori, come appunto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel tracciato della loro testimonianza e della loro lotta senza quartiere alla mafia, si è formata un'intera classe dirigente in tutti i Corpi dello Stato, che ha saputo attrezzarsi e sferrare attacchi decisivi al cuore di questa piaga; piaga che ha radici profonde e sa sempre ripresentarsi sotto spoglie diverse. Il ricordo di oggi deve avere il valore di un impegno, convinti - come siamo - che le mafie, la 'ndrangheta, la camorra e tutte le forme di criminalità organizzata, interne ed esterne, si possono arginare e battere con un'azione determinata e preventiva delle forze dell'ordine, degli apparati appositi e dello Stato, in tutte le sue articolazioni territoriali. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Li Presidente, è così: il 23 maggio del 1992 è un giorno che nessuno di noi, nessun cittadino, può dimenticare. Quella voragine nell'autostrada a Capaci, Palermo, ha creato una ferita profonda, solo in piccola parte rimarginata. È stato un evento drammatico che è entrato nel cuore della storia del nostro Paese: rappresenta una sorta di spartiacque. È stata una sferzata di consapevolezza a quanti sottovalutavano, disconoscevano, minimizzavano la portata della presenza mafiosa a Palermo, in Sicilia e nel Paese tutto. È stata una chiamata di responsabilità forte, di denuncia, per quella parte delle istituzioni e della politica che hanno creato quel sistema di collusione che ha reso Cosa nostra potente, aggressiva e capace di organizzare delle stragi: il 23 maggio a Capaci, dopo poche settimane in via d'Amelio e poi lungo il continente a Roma, a Firenze e a Milano. Giovanni Falcone un magistrato che sapeva faticare, intelligente, critico, che sopportò da più parti delle pesanti forme e tentativi di isolamento,

hanno donato la loro vita ad un Paese che se la deve meritare tutta e ciò avverrà quando avrà deciso di andare fino in fondo nell'eliminare la presenza delle mafie dalla società, dall'economia, dalla politica e dalle stesse istituzioni. Le forze dell'ordine, con passione e professionalità, la magistratura, con autonomia e intelligenza, hanno accertato le responsabilità cosiddette militari: gli esecutori materiali (chi azionò il telecomando), quelli che riempirono di tritolo il tunnel sotto l'autostrada, quelli che prepararono la strage e i capi di Cosa nostra, Riina e Provenzano, che decisero di aggredire lo Stato come mai prima di allora nella sua storia. Mancano ancora le responsabilità dei cosiddetti mandanti, di coloro che con Cosa nostra pensarono e decisero di agire, e gli eventuali intrecci di natura politica che hanno sempre caratterizzato le scelte della mafia nell'agire contro i rappresentanti delle istituzioni. Presidente, la politica deve assumersi pienamente la responsabilità di chiarire fino in fondo la natura di quelle stragi e tutte le responsabilità politico-istituzionali che ad esse sono collegate. Presidente, siamo pronti in Commissione parlamentare antimafia a donare al nostro Paese anche la più terribile, rigorosa e amara fra la politica nel contempo deve saper definire un salto di qualità come mai è avvenuto nella vita del nostro Paese. Colleghi, la lotta alla mafia deve diventare per tutti una grande priorità che deve impegnarci come mai prima d'ora, a partire dal nostro Parlamento. Diceva Giovanni Falcone: bisogna rendersi conto che la mafia è un fenomeno terribilmente serio e grave, che va combattuto non pretendendo l'eroismo di inermi cittadini, ma convergendo nella lotta le forze migliori delle istituzioni. Fino ad ora i risultati migliori li abbiamo ottenuti nella cosiddetta antimafia del giorno dopo: prima colpiscono, si riorganizzano e poi lo Stato reagisce. Dobbiamo passare a quella dimensione tanto cara a Falcone che è quella dell'antimafia del giorno prima: prevenirli, disarticolarli, scardinare il loro sistema integrato che sa agire tanto sul piano militare quanto su quello sociale, economico e politico. Oggi le proposte ci sono: dal 41-*bis* alle misure di prevenzione patrimoniale, dalla confisca dei beni al loro riutilizzo sociale e produttivo, al controllo di legalità nel sistema degli appalti, dalla lotta alle estorsioni e al riciclaggio locale e internazionale, dal sistema della compravendita dei voti financo allo scioglimento per mafia dei comuni infiltrati. Siamo ancora alle prime scelte, qui in Parlamento, al Senato; siamo ancora lontani da un'azione sistematica, profonda, in grado di sradicare il fenomeno mafioso. Molte delle proposte sono nate con Giovanni Falcone, adesso sta a noi decidere se la memoria che oggi celebriamo deve essere viva, attiva e capace di produrre risultati in grado di cancellare dal nostro Paese la presenza della mafia, o meglio delle mafie. Il Presidente della Repubblica, in un commovente intervento a Palermo, nell'aula *bunker*, di fronte a centinaia di giovani studenti, ha tracciato il cammino giusto. Le associazioni antiracket, la Confindustria siciliana, le associazioni di volontariato come Libera hanno fatto scelte positive, coraggiose ed esemplari. Adesso spetta a noi fare, fino in fondo, la nostra parte.

nel 1992, il 23 del mese di maggio, Giovanni Falcone con Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani morivano nella strage di Capaci. Una strage che diede vita ad una stagione di attacco allo Stato da parte dell'ala militare della mafia, una stagione che non esito, oggi, a distanza di 17 anni, a definire una stagione di terrorismo politico‑mafioso. Da lì sino alle stragi del 1993. E mi piace ricordare che nella notte tra oggi e domani di 16 anni fa avveniva la strage di via dei Georgofili. Giovanni Falcone, quando entrò in scena come magistrato antimafia, di fatto si trovò in una situazione di rottura di una stagione in cui lo Stato stava per cedere silenziosamente alla infiltrazione della mafia nella nostra società. Egli costruì, comprendendo fino in fondo che i fatti di mafia non potevano essere esaminati singolarmente, il lavoro dei*pool* che dovevano affrontare l'intera materia.

sino alla sentenza definitiva della Cassazione, diventando in quel modo un fatto sconvolgente nella vita del Paese e nella rottura degli equilibri. Per fare questo incontrò tanti nemici nella sua vita. caso, la fortuna di trovarmi ad essere nella sua stanza il giorno in cui otto magistrati del suo ufficio - tutti tranne uno - firmarono un documento di fiducia, perché veniva attaccato dalla politica e poi ancora attaccato e tradito da colleghi magistrati mentre doveva accedere a funzioni importanti *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Ma aveva conquistato il cuore di tanti giovani della Sicilia. È stato il primo magistrato che è riuscito a creare emozioni forti, che si sono scatenate nella società visibilmente per anni dopo la sua scomparsa.

Ovviamente tutto questo ha portato a conseguenze drammatiche, ma ha rappresentato una svolta nella vita e nella lotta alla criminalità organizzata. Cosa nostra e le sue connessioni interne ed internazionali hanno subito un durissimo colpo. Ed è vero quello che è stato detto in quest'Aula, lo dico con grande angoscia interiore. Abbiamo identificato gli esecutori materiali della strage. Abbiamo identificato - i magistrati e gli inquirenti i mandanti interni, i capi di Cosa nostra che avevano deciso l'azione, i capi di Cosa nostra di quell'epoca, che ardirono dopo le stragi si sarebbe aperta una fase in cui avrebbero trattato con lo Stato come se fossero stati un altro Stato o uno Stato nello Stato. Badate bene, stiamo parlando di cose avvenute non nel 1500, ma poco più di dieci anni fa, nella Repubblica italiana. E Giovanni Falcone aveva capito tutto questo. Per questo ha perso la vita. Io credo allora - e concludo,

tutta quella stagione, che rappresenta ancora un buco nero e buio nella storia della Repubblica italiana. Questa è la realtà di quella stagione. Restano molte cose da capire e molte da verificare; e resta da capire se il fenomeno fu tutto un fatto tra la mafia e i magistrati coraggiosi o se a questo si arrivò con tutta una serie di connessioni che sono ancora da svelare, tant'è che procure importanti stanno ancora lavorando. Credo che 17 anni siano un tempo che può consentire oggi di arrivare finalmente alla verità, perché i giovani che crescono possano sapere sempre, nel loro futuro, qual è la verità della più brutta stagione che la nostra Repubblica ha vissuto dalla sua fondazione ai giorni nostri.

ma la vita riserva a volte anche delle sorprese. Mi trovo qui oggi a commemorare Giovanni, credo che nessuno di noi possa capire la grandezza di Giovanni Falcone se non si ricorda che egli era un giudice che svolgeva esclusivamente funzioni civili, un giudice fallimentare. - riuscirono a nominare Rocco Chinnici consigliere istruttore di Palermo

Inventò, con Rocco Chinnici, un sistema di accertamento delle responsabilità penali, ma non si è mai illuso di poter risolvere il problema della mafia con i processi. I processi servivano ad accertare le responsabilità, a condannare i responsabili di fatti mafiosi,

e può anche avere addentellati all'interno delle istituzioni quando non vi è un corretto comportamento in ogni agire quotidiano, in ogni azione della vita. È solo così che la mafia può essere debellata. E Giovanni Falcone portò nell'esperienza del penale, venendo dal civile, le sue cognizioni, la sua concezione dello Stato, la sua concezione di servitore di questo Paese, insieme a Francesca Morvillo, che era del mio concorso e che è morta. Badate che la vera svolta fu impressa da quel gruppo di magistrati che iniziarono a capire la necessità di lavorare in *pool*, di lavorare senza lavorare senza il bisogno di primeggiare o di essere riconosciuti come i primi della classe. E Giovanni Falcone ha esercitato in questo modo il suo ministero durante tutta la sua vita. L'ho incontrato ancora, una settimana prima che fosse ammazzato, per la realizzazione del sogno che aveva in mente: la Direzione nazionale antimafia, ma una Direzione nazionale antimafia diversa da quella che poteva essere realizzata e che convinse il Parlamento a varare. varare. Ricordare Giovanni Falcone serve a ricordare Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, tutti gli altri, da ultimo Livatino, morti nell'adempimento del dovere, perché rappresentavano, in una terra in cui molte volte le istituzioni

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino all'11 giugno 2009. Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge collegato su sviluppo economico e processo civile, che potrebbe concludersi entro questa sera. Ricordo che per il voto finale è richiesta la presenza del numero legale. Pertanto, la seduta di sindacato ispettivo, già prevista per giovedì mattina, sarà anticipata alla seduta antimeridiana di domani, che concluderà così i lavori della settimana. Dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea in vista delle elezioni europee e amministrative, l'Aula tornerà a riunirsi martedì 9 giugno, alle ore 17, per l'esame di mozioni sulla situazione in Birmania, sugli aiuti internazionali alla salute riproduttiva e sul parto cesareo. Nel corso di tale settimana saranno inoltre discussi il disegno di legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari e il disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La calendarizzazione del disegno di legge recante disposizioni in materia dì sicurezza pubblica sarà stabilita, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni, dalla Conferenza dei Capigruppo da convocare nella giornata di martedì 9 giugno. In tale sede sarà anche previsto l'inserimento in calendario della ratifica del Trattato di Prum. Nel corso della Conferenza odierna, il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto di prevedere una prossima calendarizzazione del disegno di legge Zanda sulla riduzione del numero dei parlamentari. A tale riguardo, la Presidenza, sulla base dell'orientamento concordemente espresso dai Capigruppo, ha provveduto ad inviare una lettera al Presidente della la Commissione permanente, affinché la Commissione riprenda l'esame del complesso dei disegni di legge di riforma costituzionale sulla struttura e le funzioni delle Camere - già presentati o preannunciati - tra i quali rientra anche il predetto provvedimento di iniziativa del senatore Zanda. Ciò anche alla luce di quanto già stabilito dall'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali nella riunione del 24 marzo scorso. Presidente, lei ha riferito all'Aula quali siano state le perplessità odierne e la questione oggi sollevata dal senatore La Torre nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Vorrei fare un brevissimo *excursus*: la questione della calendarizzazione del disegno di legge del senatore Zanda sulla riduzione del numero dei parlamentari

del senatore Zanda, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, si svolgerà congiuntamente a quello di altre proposte di revisione costituzionale in materia di struttura e funzione delle Camere, già presentate o preannunciate.

Fino a quando essi non verranno calendarizzati in Aula noi solleveremo la questione. Peraltro, se si tratta di una questione così rilevante per il Gruppo del Partito Democratico, non credo sia meno rilevante per il Popolo della Libertà, atteso che addirittura il Presidente del Consiglio pensa di ricorrere ad una legge di iniziativa popolare e di raccogliere le firme, con qualche dispendio di tempo, per discutere esattamente di quanto è già presente in Parlamento, è già all'attenzione dei parlamentari e, come ricorderanno i colleghi, sia pure *sub specie*

benissimo calendarizzare tale provvedimento, ovviamente ove concluso in Commissione (nessuno vuole una lettura approssimativa). Poiché ne discutiamo da

tratta di una questione politica preliminare, signor Presidente. Lei sa quali sono i rapporti che il Gruppo del Partito Democratico sempre in Conferenza dei Capigruppo ha teso a mantenere con i colleghi e soprattutto con lei, ma non voteremo più nessun calendario fino a quando la questione non verrà posta all'ordine del giorno dell'Aula.

Signor Presidente, prendiamo atto che finalmente in Parlamento c'è la volontà di tutti di ridurre il numero dei parlamentari, cosa che la Lega ha sempre sostenuto.

dal Gruppo PD)*, visto che l'unica riforma della Costituzione che è stata votata in Parlamento nella storia di questa Repubblica è stata poi bocciata da un *referendum* popolare

Siamo contenti che ci sia questa richiesta da parte di tutto il Parlamento, dai colleghi del Popolo della Libertà, dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico. Dunque, ritengo sia giusto arrivare ad una calendarizzazione di queste riforme tenendo conto che devono essere discusse anche con le altre riforme istituzionali, sempre all'attenzione della 1a Commissione, che tutti vogliono, o almeno hanno sempre dichiarato di volere: mi riferisco alla fine del bicameralismo perfetto e dunque all'istituzione

parte del programma elettorale presentato dalla Lega e dal Popolo della libertà durante le elezioni e che la garanzia che andremo a cambiare questo Paese ce l'abbiamo nella figura di Umberto Bossi, ministro delle riforme di questo Governo *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal già votato il federalismo fiscale insieme in quest'Aula, parlando e dialogando con tutti ed è quanto vorremmo fare anche con queste riforme. Presidente, colleghi il Gruppo dell'Italia dei Valori nota con grande piacere che siamo tutti interessati ad una riforma che diminuisca il numero dei parlamentari. Questo può rassicurare quell'alta carica dello Stato che voleva ricorrere direttamente al popolo per fare non si sa che sotto il profilo costituzionale. Il Parlamento è nelle condizioni di esaminare il provvedimento e di farlo a breve. Noi accettiamo la sfida e vogliamo che venga accelerato attraverso una tempestiva calendarizzazione dei lavori. tal proposito, è vero che venne approvata una riforma qualche anno fa. Ricordo che quella riforma rinviava, se non erro, al 2016 la riduzione dei parlamentari - una riforma "a babbo morto" - e non riguardava soltanto

Oggi abbiamo la possibilità e la volontà di farlo. Sappiamo che la riduzione dei parlamentari è inserita in un più complessivo sistema di riforme della nostra Costituzione. Accettiamo la sfida del Presidente del Consiglio e anzi la rilanciamo,

del successivo *referendum* confermativo, chiesto - come le norme della Costituzione consentono - dalla

Insieme ad un Parlamento più efficiente e più snello, serve un Governo che abbia maggiori poteri, serve una revisione del bicameralismo. Noi abbiamo una visione globale, complessiva e seria della riforma della Costituzione e delle istituzioni, a differenza vostra, che su questi temi avete fatto sempre un sostanziale ostruzionismo. Non vedo poi quale meraviglia dovrebbe suscitare

ma un partito politico può ben promuovere nel Paese, *a latere* e non in alternativa, proposte di iniziativa popolare, per dare più forza e consenso ad una scelta di cambiamento. E mi pare paradossale che riteniate questa via non percorribile. *(Commenti dal che proprio la Commissione affari costituzionali nei prossimi giorni ascolterà perfino Beppe Grillo che, pur non avendo un partito e pur non sapendo quanti voti rappresenta,

ma anche di una più ampia riforma delle istituzioni, perché la seconda parte della Costituzione ha bisogno di essere rivista. Ci auguriamo di incontrarvi su questa strada e che non rimaniate ancorati ad una visione un po' passatista, in modo che il Parlamento possa autoriformarsi. E che non facciate poi i *referendum* per mantenere il numero di poltrone inalterato, come avete già fatto.

Signor Presidente, siamo alla quarta lettura di un provvedimento che sposa la riforma del processo civile con interventi di sviluppo economico per dar vita ad un sistema giudiziario efficiente che dispensi certezza giuridica e promuova lo sviluppo economico e il benessere. È noto a tutti che una giustizia civile e rapida fa girare velocemente l'economia e l'obiettivo principale che questo provvedimento, appunto, persegue è la riduzione dei tempi del processo, che oggi sono drammaticamente lunghi e collocano l'Italia nelle graduatorie internazionali sull'efficienza dietro ad alcuni Paesi africani. come tutti gli interventi riformatori anche questo ha sollevato dei distinguo, ma tutto si può dire tranne che la situazione poteva essere lasciata così com'è. Ci sono provvedimenti dal lato della domanda di giustizia - penso al principio di lealtà processuale - per responsabilizzare l'iniziativa degli avvocati, proprio tenendo conto della litigiosità che caratterizza e connota il nostro sistema, senatore D'Ambrosio. Ci sono poi provvedimenti anche dal lato dell'offerta, volti alla riduzione dei tempi processuali, alla semplificazione dei riti, alla mediazione, proprio per diminuire il pesante di Stato per la giustizia*). Ma consentitemi solo di soffermarmi brevemente sul filtro in Cassazione. Si tratta di un'innovazione assai importante, sostanziale, significativa, questa sua importanza è stata sottolineata in un recente studio proprio dalla Banca d'Italia. Ebbene, questo studio, basato sulla letteratura economica, segnala che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'efficienza dell'ultimo grado di giudizio, perché condiziona le scelte delle parti e il comportamento dei giudici nei precedenti gradi di giudizio. È normale - e lo dico al senatore Delogu che questa mattina ha introdotto il tema del filtro in Cassazione - che una norma come quella attuale, che presenta che presenta profili di assoluta novità, possa determinare discussioni, approfondimenti, dibattiti che possono portare, come è stato, a rivisitazioni della formulazione del testo originario. Questo è proprio il cuore della dialettica parlamentare. La norma approvata dalla Camera dei deputati, e all'unanimità, cioè con l'approvazione della maggioranza e dell'opposizione (e credo, quindi, che questo non possa essere considerato uno scempio, come ha il senatore Li Gotti), introduce un significativo mutamento di prospettiva rispetto alla disposizione approvata in seconda lettura dal Senato. In base a questo testo - forse è bene spiegarlo ancora una volta - la Corte di cassazione sarà chiamata a verificare se sussista una causa di inammissibilità del ricorso. Si è cambiata quindi la prospettiva: prima si dichiarava che il ricorso era ammissibile, mentre oggi si afferma che il ricorso in linea di principio è ammissibile, salvo che ricorra una delle cause di inammissibilità previste dell'articolo 360-*bis* del codice. Il testo approvato dal Senato in seconda lettura è andato incontro ad alcune osservazioni critiche, in quanto la norma sul filtro in Cassazione attribuiva alla Corte un potere eccessivo riferimento

«di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento». Dunque, si tratta di un potere discrezionale che è stato ritenuto troppo ampio. Il testo approvato dalla Camera aggancia invece la valutazione di inammissibilità del ricorso al verificarsi di presupposti oggettivi. Anche nella nuova formulazione, la norma sul filtro consente alla Corte di cassazione di esaminare il ricorso nel merito quando, in base all'esame dei motivi di ricorso, emerge la necessità di confermare o mutare l'orientamento della Corte. Si tratta di una norma,

gli interventi predisposti sono mirati a ridare mobilità e respiro ad un sistema gravemente compromesso, a deflazionare il terribile carico di arretrato

«La 1a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.1, sulla quale il parere è di semplice contrarietà».

Signora Presidente, il parere del Governo va nello stesso senso del relatore, tenendo conto che siamo alla quarta lettura del provvedimento. Quindi, invito caldamente i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti, il parere sarà contrario su questi come sugli altri

tutti ricadono sotto la competenza del Ministero dello sviluppo economico. È pertanto giusto, a mio avviso, che il Governo inserisca, per il buon funzionamento dell'ASI, un nessuno è designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;

di avere un membro designato anche dal Ministro dello sviluppo economico nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana. italiana. La seconda parte dell'ordine del giorno, invece, tiene conto di due argomenti importanti: in primo luogo, le tecnologie nel settore aeronautico e spaziale ormai sono estremamente similari, quindi c'è una sinergia molto forte in quel contesto

basti pensare alle telecomunicazioni spaziali, alla navigazione spaziale per quanto riguarda i trasporti, ai problemi relativi all'ambiente e all'osservazione della terra, per quanto riguarda

chiedono la stessa cosa, e cioè l'inserimento nel Consiglio di amministrazione dell'ASI di un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico, sarebbe opportuno avere in entrambi la stessa enunciazione. Credo sia più opportuna quella del G27.1, in quanto l'espressione «ad adoperarsi» mi sembra più appropriata rispetto a «prevedere», visto che per prevedere effettivamente una diversa composizione di questo

Ricordiamo tutti le recenti problematiche che sono derivate dall'assenza di una disciplina specifica e che si sono manifestate anche in relazione alle ultime elezioni politiche con il ricorso dell'onorevole Pizza contro il provvedimento di esclusione della sua lista dalle ultime competizioni elettorali: ciò, oltre a produrre dei forti contrasti giurisprudenziali, ha rischiato di compromettere addirittura lo svolgimento delle elezioni politiche del 2008. Noi condividiamo la scelta che è stata compiuta al comma 2, lettera *d*) dell'articolo 44, di tipizzare un procedimento *ad hoc* per le controversie concernenti atti di procedimenti elettorali preparatori per le elezioni del rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Non possiamo però assolutamente condividere l'attribuzione di queste controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

con le quali è stata censurata l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla base del parametro utilizzato anche in questo caso dei blocchi per materie. materie. In questo senso, abbiamo presentato gli emendamenti 44.1 e 44.300, volti appunto a modificare questa situazione.

di arrivare all'approvazione definitiva

Dichiaro aperta la votazione.

Cassazione, accogliendo finalmente la nostra proposta e parlando di ricorso «inammissibile» invece che «ammissibile». Peraltro, per un refuso, è rimasta è rimasta una impostazione letterale sbagliata secondo la logica della lingua italiana e secondo il diritto. Si tratta della parte che concerne il riferimento all'esame dei motivi che non offre elementi «per confermare o mutare» l'orientamento della Corte di cassazione.

chiamare - noi ci dissociamo. I giuristi e gli esperti di diritto se la prenderanno con chi ha chiuso un occhio e accettato errori così banali.

Camera. All'articolo 51, leggendo il Resoconto della Camera dei deputati, non è chiaro il passaggio dal rito sommario a quello ordinario. C'è un punto oscuro che forse il Governo dovrebbe chiarire, anche nell'ambito della delega che gli è stata conferita per il procedimento di unificazione in relazione proprio al rito sommario. Si legge che ai fini dell'introduzione del procedimento sommario, la parte convenuta ha soli 10 giorni di tempo prima dell'udienza per costituirsi. Ove mai il giudice, come prevede la norma, non ritenesse che quella causa debba essere trattata con rito sommario, la disposizione prevede che si fissi l'udienza, ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile. Quello che invece la norma non prevede, e su cui chiedo chiarimenti, è che nel fissare l'udienza si rimettano i termini alle parti al fine di preservarle dalla decadenza. Per chiarezza della norma ritenevo utile questo intervento e ringrazierei il Governo se replicasse.

dell'articolo 51 è assai chiara in quanto recita testualmente che il giudice, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria,

la prima udienza del procedimento di cognizione ordinaria, nella quale le parti possono chiedere, in base al comma sesto del medesimo articolo 183, le memorie istruttorie. Quindi non c'è alcun bisogno di fissare ulteriori termini, al di là del rinvio all'articolo 183, perché quest'ultimo già prevede la possibilità per le parti di chiedere le memorie necessarie per una istruttoria completa.

dal Senato, non viene posto in votazione in quanto le modifiche al testo ivi recate consistono in un mero coordinamento numerico, reso necessario dalla soppressione di un precedente articolo.

Onorevoli colleghi, di fronte all'ennesimo, tragico incidente sul lavoro, cui hanno perso la vita tre operai, in Sardegna, questa Presidenza vuole esprimere il sentimento più forte di preoccupazione e dolore per le vittime e i loro familiari. La civiltà di un Paese è anche civiltà del lavoro. Il diritto alla vita e alla salute non può essere compresso da nessun'altra logica. Questi episodi non possono, non devono più accadere. Lo dobbiamo ai cittadini, alle famiglie, a tutti i lavoratori. Vi invito, in segno di lutto, ad osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, vorrei che quest'Aula ascoltasse i nomi delle tre persone scomparse:

delle cosiddette aziende d'appalto della Saras, che ha una grande raffineria a Sarroch, vicino Cagliari. Lì sono morti, dentro una cisterna di gasolio che evidentemente doveva essere pronta per la manutenzione, ma che era invece piena di azoto; sono rimasti soffocati, in una gara di solidarietà, l'uno cercando di salvare l'altro. Apprezzo la presenza in Aula del ministro Sacconi e chiedo che il Governo riferisca prima possibile all'Aula su quanto

Il Parlamento sia il più possibile attento a non compiere passi falsi, a non fare riforme affrettate, a considerare con il massimo realismo cos'è il lavoro in Italia e cosa sono i lavori, non solo quelli dei lavoratori dipendenti tutelati, ma anche quelli che dipendono dalle commesse a cascata, di un sistema industriale che cerca di risparmiare in ogni modo. Signor Presidente, quando si legge che sono morti in un incidente sul lavoro due ragazzi di 26 e 27 anni e un signore, padre di tre figli, è veramente difficile trovare le parole per dire qualcosa che vada oltre la commozione più profonda. Sono morti nello stabilimento della Saras, a pochi chilometri da Cagliari,

Come Gruppo Lega Nord ci associamo al sentimento di cordoglio per queste notizie che non vorremmo mai e poi mai apprendere: notizie di lavoratori che muoiono.

Sapete quanto sono legato alla terra sarda, al popolo sardo, per le mie origini e per il sangue che mi scorre nelle vene. Quindi, è veramente un momento di grande cordoglio per tutti noi.

In ogni caso un lavoratore che muore è un lavoratore che ha perso la vita mentre stava esercitando un diritto costituzionale. Questa è l'ennesima tragedia che colpisce la nostra Italia e i nostri lavoratori. Ma credo che ci troviamo in un momento importante in cui il Governo con il decreto correttivo sul testo unico sulla sicurezza sta portando

saremo vigili affinché il testo unico sulla sicurezza continui ad essere uno strumento per la tutela dei lavoratori e non venga stravolto. È importantissimo che queste norme siano efficaci,

anche la Commissione d'inchiesta sulle morti bianche sicuramente si attiverà in modo deciso e determinato perché la legislazione, i controlli e gli strumenti per tutelare i lavoratori siano sempre più efficaci.

purtroppo sta colpendo troppo frequentemente tanti altri lavoratori. Se fate attenzione, la stragrande maggioranza delle morti sul lavoro si stanno verificando soprattutto

Come è noto, una situazione lavorativa come quella in discussione è oggetto della vigilanza e delle attività ispettive del Servizio sanitario regionale. con ogni probabilità, ci troviamo di fronte ad un contesto lavorativo ragionevolmente sottoposto ad un adeguato controllo, non solo istituzionale, ma anche di tipo sociale, date le caratteristiche

a partire dalla responsabilità delle imprese. Occorre mettere la persona nelle condizioni di essere fino in fondo cosciente e consapevole di tutti gli elementi che possono determinare pericolo per la sua incolumità, in modo da prevenire esiti letali come quelli che si sono in questo caso prodotti. Pertanto, mi unisco alle considerazioni che si sono svolte e a quelle che sollecitano un'attenta ponderazione delle modifiche che sono state ipotizzate al decreto contenente il testo unico, perché le morti sul lavoro non possono non toccare le coscienze di tutti, nella ricerca di soluzioni quanto più effettive.

non c'è dubbio che vi è la massima necessità di riformare il processo civile e rendere più efficiente la macchina amministrativa, nonché trovare urgenti misure per uscire dalla crisi economica. Ci tengo a ricordare la classifica internazionale sui tempi processuali, contenuta nel rapporto *Doing

Quanto ad efficienza della giustizia, il nostro Paese viene addirittura dopo l'Angola, il Gabon, la Guinea e Sao Tomé. Questi dati, signora Presidente, hanno suscitato lo sconcerto maggiore alla fine dello scorso gennaio, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, a giustificazione degli allarmi lanciati a ripetizione dal Consiglio d'Europa.

Basti pensare che nel 2008 lo Stato ha dovuto pagare ai cittadini più di 32 milioni di euro di risarcimento per danni legati al protrarsi dei processi. Tornando al provvedimento in esame, non ci trova d'accordo la decisione del Governo di intervenire in modo parziale attraverso un provvedimento *omnibus*. Ciò ha purtroppo pregiudicato il confronto parlamentare con ripercussioni negative sulla qualità delle norme e sulla coerenza dell'ordinamento. che nel tortuoso tragitto dalla Camera al Senato e poi dal Senato alla Camera, il provvedimento ha riportato l'aggiunta di numerosi nuovi articoli e ulteriori deleghe.

la prova testimoniale, che poteva essere meglio definita, la mini riforma del processo civile, che avrebbe dovuto introdurre norme più utili per l'efficienza della giustizia e la riduzione dei tempi processuali precedentemente indicati, tenendo conto anche del fatto che la lentezza dei processi in Italia è stata causa di 51 delle 82 condanne inflitte dalla Corte europea di

In parte le risorse finanziarie vengono acquisite attraverso i fondi FAS, i fondi per le aree sottoutilizzate, impiegati non per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate ma per le più diverse ragioni. In questo modo il processo di sviluppo delle imprese e dei territori viene fortemente depotenziato. Un'altra fonte è quella degli interventi strutturali di politica economica e delle riduzioni lineari delle autorizzazioni di spesa, ma tutto nell'ambito di una preoccupante incertezza di collocazione effettiva dei fondi. Con riferimento

meno indebitate rispetto ad altri Paesi sviluppati. Lo stesso vale per le nostre imprese. Possiamo pertanto puntare su un elemento molto importante, la tenuta della domanda interna, grazie a questa propensione dei nostri cittadini e delle nostre imprese. La difficoltà, però, per il nostro Paese sta nel fatto che anche la nostra economia dipende dall'*export*, cento del prodotto interno lordo, anche se naturalmente meno della locomotiva europea delle esportazioni, cioè la Germania, con il 48

e sotto il profilo delle piccole innovazioni in materia di giustizia esso risente di improvvisazione e della mancanza di un quadro chiaro di riferimento. Mi dispiace molto di questo perché il codice civile non dovrebbe essere una normativa

ha presentato una serie di proposte migliorative tutte ispirate dal rifiuto di una posizione pregiudiziale e dalla ricerca delle politiche più utili per il Paese. quali la semplificazione normativa, che è necessaria ma talvolta è realizzata in modo davvero complicato, la pubblica amministrazione, la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, la Conferenza dei servizi: tutto questo nella convinzione che la pubblica amministrazione debba tornare ad essere vista non solo come un vincolo o come un impaccio, ma anche come una grande risorsa per le politiche pubbliche nazionali e che che il procedimento amministrativo debba tornare ad essere, anche sotto il profilo della cultura giuridica ed istituzionale, quello che è stato, cioè un grande strumento di mediazione sociale che consente partecipazione dei cittadini, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. È stato anche affrontato in modo insufficiente il tema del turismo e del consiglio d'amministrazione dell'ENIT. Siamo tutti molto convinti che il turismo meriti una politica molto intensa perché è una delle risorse primarie per tutto per tutto il nostro Paese e per le varie Regioni che lo compongono. Giudichiamo invece con favore la creazione di organismi di conciliazione previsti dal provvedimento. Ma non è stato definito in modo chiaro e netto l'impatto di queste norme nella modifica del processo civile, il che ci lascia ovviamente perplessi. Abbiamo assistito al conferimento di ulteriori deleghe sulla base delle previsioni Le famiglie e le imprese si trovano in grande difficoltà. Sono loro la risorsa più importante per far ripartire l'economia ed il consumo. La risposta a questo riguardo, purtroppo, non è del tutto soddisfacente. Per questo il Gruppo UDC, SVP e Autonomie si asterrà dal voto finale su questo disegno di legge. Si tratta di una posizione assunta in modo convinto e con la quale, nonostante tante perplessità, vogliamo apprezzare gli sforzi compiuti e dare il nostro contributo allo sviluppo del Paese.

peggiorata dalla Camera dei deputati, peggioramento al quale noi abbiamo assistito con una grande rassegnazione, pur se questo stesso peggioramento era stato condiviso dalla maggioranza. Ricordo che in Commissione giustizia proprio il senatore Berselli, Presidente di tale Commissione, aveva rilevato un peggioramento del testo, la necessità di intervenire per modificarlo e consegnare al Paese e ai cittadini un testo quanto meno efficace nelle norme modificate. Invece, la logica della politica si sostituisce

la malattia del sistema giustizia, nel senso che una giustizia che non funziona incide anche sull'economia, perché impedisce e comunque non invoglia investimenti nel nostro Paese e non dà risposte alle domande di riparazione, di restituzione, di riconoscimento dei diritti. Si tratta di un fatto al quale stiamo assistendo da troppi anni. Perché questa regressione? Perché stiamo andando sempre più pesantemente indietro? Perché non riusciamo a raddrizzare a raddrizzare la schiena e ad affrontare i problemi come essi meritano? Sapete che nel giro dei prossimi tre anni, a cominciare da quello corrente, i tagli di

il personale amministrativo della giustizia è già carente di oltre 8.000 unità? Ogni anno, a causa del *turn over*

Stanno scomparendo i cancellieri, figura centrale per la celebrazione delle udienze e per l'attività di assistenza al magistrato. magistrato. Tagli del personale e di risorse, un timido accenno di riforma del processo civile, ma non accompagnato da una seria volontà...

che il nostro sistema ed anche la formazione culturale di noi che operiamo nel mondo della giustizia si siano modulati sulla patologia del processo, sicché ci sentiremmo smarriti il giorno in cui il sistema giustizia in Italia dovesse cominciare a funzionare; non sapremmo più come gestire qualcosa che funziona, perché ormai siamo attrezzati a gestire qualcosa che non funziona. Questa è la resa che stiamo cogliendo nel Paese: un'accettazione, senza alcuna reazione effettiva, della patologia che affligge il sistema; è l'aspetto più negativo, nel senso che non penso che si abbia a cuore veramente il tema della giustizia nell'agenda di questo Governo. I progetti avviati, pur materia di discussioni approfondite che avevano coinvolto maggioranza ed opposizione, con una visione unitaria del progetto di riforma del processo civile nella scorsa legislatura, con voto unitario in Commissione giustizia del Senato, vengono abbandonati e non coltivati dal Governo e dalla maggioranza. Per quale motivo?

Penso che la politica dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire se veramente questo settore è per noi ritenuto essenziale, sicché necessita di interventi radicali, decisi e ragionati ma efficaci, oppure se si vuole intervenire con *spot* propagandistici quali: riformiamo la giustizia, da domani i cittadini avranno una giustizia più veloce, tutti saranno soddisfatti e finalmente il processo civile italiano funzionerà. da domani tutto questo non avverrà nel modo più assoluto sicché noi, se riusciamo ad abbandonare la politica dello *slogan* e dello *spot* e con umiltà ci chiniamo sui problemi, li valutiamo, ci confrontiamo e quando lo facciamo molte divisioni cadono. Questa è l'amarezza che riscontriamo. Quando ci confrontiamo ragionando sui problemi nelle Commissioni, cadono le divisioni ideologiche e partitiche. Si ragiona seriamente. Poi arriva il virus di questa cattiva gestione della politica che annulla tutte le buone volontà. Questo è il risultato della cattiva volontà. Noi non votiamo e non accettiamo questo risultato perché vogliamo ancora sperare che attraverso il dialogo, il confronto, la lealtà la stima che esistono nei rapporti tra noi nell'ambito dei luoghi in cui lavoriamo potremo ottenere ad un risultato serio e convincente. Nella fiducia e nella speranza che questo possa accadere, noi diciamo un no convinto a questa cosiddetta riforma che è solo una battaglia di retroguardia ed è solo uno *spot* propagandistico.

Noi ragioniamo in termini diversi e, poiché siamo anche in un momento di congiuntura tanto difficile, riteniamo che qualsiasi cosa che va in senso migliorativo vada accolta a braccia aperte e con estrema fiducia.

parzialmente sulla riforma della pubblica amministrazione ed altrettanto parzialmente sulla riforma della giustizia. Sappiamo quanto ci sia bisogno

il solo preannunciare che ci saranno e verranno esposti e resi pubblici i tassi di presenza o di assenza nelle pubbliche amministrazioni ha già giovato: soltanto l'annuncio ha già prodotto risultati concreti. La domanda di giustizia che percepiamo dal sistema delle imprese e dei cittadini è enorme: come facciamo a fare orecchie da mercante, a fare i sordi? Cosa avremo domani, approvata questa riforma? Anzitutto una giustizia più civile, più rapida, efficace e snella;

notaste un dato: ormai non c'è più un imprenditore, un artigiano, un commerciante che non si renda conto di quanto sia indispensabile disporre di una giustizia civile che funziona, proprio in ragione della competitività, che poi ricade sulla propria attività. Già il collega Peterlini della Volkspartei ha fatto un piccolo quadro della situazione: 5 milioni di cause pendenti. Questa è la fotografia del nostro Paese: quasi 1.000 giorni per definire un causa in primo grado; più di 1.500 per definirla in appello.

Torniamo allora agli aspetti economici. Per recuperare un credito di una disputa commerciale in Italia servono 1.210 giorni; 300 circa in Germania, poco più di 300 in Francia (e siamo sugli stessi standard in Giappone). dati, riusciamo a capire quanto sia difficile fare impresa nel nostro Paese. Il pacchetto degli interventi

abbreviate e semplificate e, infine, a garantire il diritto ad avere una sentenza certa in tempi ragionevoli. È aumentata la competenza per valore del giudice di pace. Sappiamo quanto sia indispensabile oggi la magistratura onoraria per l'amministrazione della giustizia e crediamo che questa figura vada ulteriormente qualificata, anche perché è l'unica in grado di decongestionare e liberare i giudici togati da una grande mole di cause. Si è semplificata la decisione della lite con tempi certi per ogni singola attività processuale. È stato introdotto il nuovo istituto della prova testimoniale scritta e ci accorgeremo subito di quale funzione acceleratrice produrrà. Oggi abbiamo migliaia di lavoratori, migliaia di artigiani e piccoli imprenditori che perdono intere giornate di lavoro soltanto per andare davanti ad un giudice a confermare di aver emesso una fattura o una ricevuta fiscale.

Si è poi fatta una semplificazione storica dei riti. Oggi abbiamo circa 30 riti. Con la delega che stiamo dando al Governo avremo soltanto tre riti processuali: il rito del lavoro, l'ordinario di cognizione ed il sommario di cognizione. Tutto il resto sarà eliminato. Otterremo più certezza, più chiarezza e più tempestività, in sostanza la vera tutela dei diritti di tutti i cittadini. Sarà incentivata la conciliazione, un grandissimo strumento (di cui continuiamo a parlare, ma poi vediamo con che fatica lo si approccia) che consentirà una giustizia estremamente rapida

sicuramente una giustizia molto più efficiente. D'altronde, per entrare in questo Governo, una delle grandi questioni

*(PD)*. Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, anche in questa quarta lettura del provvedimento oggi all'esame del Senato, il Partito Democratico deve esprimere le proprie valutazioni negative. Già in seconda lettura, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, il senatore Zanda aveva segnalato le nostre fortissime perplessità in ordine ad un disegno di legge nato per lo sviluppo economico del nostro Paese, ma ben presto dirottato verso altre materie e altri settori (la semplificazione, il processo amministrativo, il procedimento elettorale, le rappresentanze consolari, la Corte dei conti, una miniriforma del processo civile, una proroga della proroga in materia ambientale, la Carta nazionale dei servizi e via dicendo). Il tutto, per di più, accompagnato dalla previsione di norme delega al Governo a raffica (quattro deleghe nel testo originario e altre cinque contenute in emendamenti presentati e approvati in seconda lettura dalla maggioranza) tra l'altro, senza il rispetto dei dettami di rango costituzionale, relativi alle necessità di determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi e di indicazione di oggetti ben definiti, come imposto dall'articolo 76 della Costituzione. Inoltre, la presentazione, tra una lettura e l'altra, di decine e decine di emendamenti, ad opera di Governo e maggioranza, dà perfettamente il senso di un testo di legge improvvisato nel suo disegno iniziale, raffazzonato nel suo procedere e articolarsi

di volta in volta, nuove norme, per correggere, emendare e cercare di completare. Quel che ne è uscito, a ben vedere, non può che lasciarci assolutamente insoddisfatti, tutto in quanto i gravi problemi di metodo da noi ripetutamente segnalati, anche oggi in quest'Aula, dal senatore Galperti e dalla senatrice Incostante, ci impongono di rinnovare la nostra critica di fondo, a causa dell'abuso da parte della maggioranza e del Governo della decretazione d'urgenza, dei maxiemendamenti e di deleghe per lo più in banco, oltre che incostituzionali: quindi, politicamente non accettabili. Addirittura in materia ambientale si prevedono deleghe primarie e correttive, si fanno le deleghe delle deleghe, deleghe interpretative e correttive che tagliano fuori il Parlamento e le sue Commissioni di merito. Mi torna in mente, a questo proposito, la critica formulata circa dodici anni fa dall'allora capo dell'opposizione parlamentare che, criticando le troppe deleghe al Governo di allora (34), parlò di espropriazione del Parlamento e di rischio per la democrazia. Quel capo dell'opposizione - guarda un po' - era l'onorevole Berlusconi e, se non smentisce anche quelle dichiarazioni riportate allora da «Il Sole 24 Ore», mi domando cosa dovrebbe dire ora del suo Governo, che in un anno si è già fatto attribuire 46 deleghe. Tutto ciò, e non solo questo, ci fa parlare di una grave degenerazione in atto nei rapporti tra Parlamento e Governo, nonché nel doveroso equilibrio tra poteri dello Stato, fondamento della nostra democrazia parlamentare. Se poi scendiamo nello specifico del disegno di legge, ci rendiamo conto di come si tratti, particolarmente per il variegato settore della giustizia amministrativa e civile, di interventi disarmonici, quasi casuali, con deleghe a catena che affidano a future ed imprevedibili decisioni del Governo e degli uffici amministrativi ministeriali questioni delicatissime che attengono ai diritti civili e all'esercizio della giurisdizione (anche quella di controllo), su cui invece dovrebbero istituzionalmente essere assolutamente prevalenti l'attività, la valutazione e la decisione del Parlamento. La miniriforma in materia processual-civilistica è estremamente emblematica a questo proposito. Nella passata legislatura si era arrivati congiuntamente, maggioranza ed opposizione, alla predisposizione di un testo di vera riforma del processo civile, approfondita e completa, auspicata da tutti: avvocatura, magistratura e studiosi del diritto. Quel testo, condiviso sostanzialmente da tutti, è stato ripresentato in questa legislatura dal Partito Democratico, ma, forse soltanto perché lo ha presentato il Partito Democratico, ora è stato rifiutato dal Governo che diceva di aver fretta e di voler intervenire rapidamente, non preoccupandosi nemmeno delle osservazioni e delle proposte della sua stessa maggioranza in Senato. È stato così trasmesso per la terza lettura alla Camera dei deputati un testo gravemente monco, a causa soprattutto del rifiuto del Ministro della giustizia di accogliere le nostre proposte. Alla Camera dei deputati, pressati da avvocatura e magistratura, ma specialmente dall'irrazionalità di alcune disposizioni approvate in quest'Aula, maggioranza e Governo hanno accettato di por mano ad un minimo di emendamenti sollecitati dai nostri colleghi del Partito Democratico, con particolare riferimento al cosiddetto filtro in Cassazione. Ora, il testo è tornato con queste modifiche dopo un viaggio troppo lungo e tortuoso, che si sarebbe potuto evitare se solo si fossero volute raccogliere le sollecitazioni del nostro Gruppo. Non si tratta ancora di una riforma del processo civile, ma qualche piccolo passo avanti è stato fatto, pur tra rinnovate proteste e contestazioni, anche oggi, da parte - nello specifico - dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana. Quello che però non è assolutamente accettabile sono la protervia e l'arroganza con cui il Governo procede in questa materia, perché anche di fronte ad errori evidenti, come è emerso dall'illustrazione odierna dei nostri emendamenti, tira diritto per la sua strada, incurante delle preoccupazioni istituzionali dell'opposizione. Soprattutto, di fronte alle esigenze di giustizia del cittadino comune (esigenze urgenti), il Governo sceglie di non trattare alcune parti del processo civile, prima fra tutte la fase esecutiva, all'evidenza una delle più bisognevoli di interventi urgenti proprio nell'ottica di una certezza del diritto ed effettività delle decisioni giurisdizionali; inoltre, il Governo privilegia, per altro verso, di farsi destinatario di numerose deleghe. motivi, di istituti innovativi e di interventi urgenti si discuterà tra anni e anni: penso alla delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei riti, ovvero in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero ancora alla delega per il riassetto del processo amministrativo, così come in tema di digitalizzazione e informatizzazione del processo civile. Alla faccia della vostra tanto conclamata propaganda sulla necessità di accelerare i processi. Se poi si considera la predilezione di questo Governo per le deleghe, anche in materia di processo penale (ad esempio in tema di notificazioni o di sospensione del processo *in* *absentia* o di digitalizzazione e informatizzazione del processo penale o di elezione dei vice procuratori onorari o di misure cautelari disposte dal tribunale collegiale), si ha la netta sensazione di una volontà di allontanare nel tempo la soluzione di problemi concreti ed urgenti e di estromettere il Parlamento da decisioni delicate in materia di diritti civili, di giustizia e di controlli sulla pubblica amministrazione, per non recar noia al manovratore o per poter meglio gestire l'intera materia secondo scelte e criteri non esplicitati, sotterranei e comunque ambigui. Il Partito Democratico non può accettare questo comportamento gravemente lesivo, più che delle prerogative dei singoli parlamentari o dei singoli magistrati, dei princìpi fondamentali che regolamentano i rapporti tra poteri dello Stato, princìpi che stanno alla base del nostro ordinamento democratico e della nostra Repubblica, princìpi trasparenti, che sono espressione della volontà popolare, il cui massimo organismo di rappresentanza è costituito dal Parlamento (minoranza ed opposizione insieme);

svillaneggiato o addirittura menomato dal comportamento del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio dei ministri. Per questi motivi, il Partito Democratico voterà contro questo disegno di legge.

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che quest'oggi l'Aula del Senato si appresta ad approvare torna da noi dopo una terza lettura alla Camera dei deputati, con modifiche peraltro ‑ è bene dirlo ‑ largamente di dettaglio, perché un approfondito lavoro è stato svolto in questo ramo del Parlamento. questo aspetto proprio per sottolineare quanto è stato fatto, accogliendo numerose proposte emendative, provenienti in particolar modo dall'opposizione.

Esiste infatti un nesso inscindibile tra sviluppo economico, semplificazione amministrativa e riforma dei processi civile ed amministrativo, tra di loro necessariamente connessi. già presente nel Documento di programmazione economico‑finanziaria, laddove la riforma, in particolare del processo civile (che però necessariamente si doveva accompagnare, quanto meno *in* *nuce*, a quella del diritto amministrativo), venne appunto individuata come uno dei fattori di sviluppo economico del Paese.

ma il mantenimento delle sole leggi utili e adeguate ai tempi, di chiara interpretazione, di facile e immediata applicabilità, sia da parte della pubblica amministrazione (il cui funzionamento nei confronti degli utenti

Questa è, onorevoli colleghi, la direzione nella quale siamo andati. Abbiamo dettato nuove regole per la redazione dei testi normativi, che finalmente li rendono comprensibili in ciò che abrogano, in ciò che disciplinano e nei loro rinvii normativi. Abbiamo tempi certi e*iter* semplificati per i procedimenti amministrativi. Abbiamo razionalizzato i flussi finanziari e i fondi strutturali per le aree sottosviluppate (uno dei fattori principali per il recupero della competitività economica del Paese). destinato particolare attenzione (attraverso l'istituzione di un apposito fondo) ad uno dei settori vitali dell'economia nazionale, quello del turismo. Abbiamo adeguato le reti di comunicazione pubblica e privata, soprattutto nelle aree sottosviluppate. delegato il Governo - sì, perché la tempistica è tale per cui non sarebbe stato possibile farlo immediatamente, ma questo processo andava necessariamente avviato - ad adottare una riforma del processo amministrativo, introducendo però intanto una prima norma di civiltà e di equità: l'equiparazione del regime delle sanatorie, delle nullità e delle notificazioni fra processo civile e processo amministrativo. Già con questo abbiamo adottato un primo passaggio semplificatore e di chiarezza, affrontando al cuore del problema la parte più necrotica di questo grande malato che è la giustizia civile la fase contenziosa, quella della più alta tutela dei diritti - con una riforma di realismo e di buon senso. Bene ha fatto il collega Divina a ricordarlo, perché nessuna delle norme che abbiamo adottato è stata contestata nel merito, né sarebbe stato possibile farlo. Ed è un primo significativo passo in avanti. Forse potrà essere essere semplicisticamente la logica del bicchiere mezzo pieno. Ebbene, noi plaudiamo alla logica del bicchiere mezzo pieno rispetto al nulla assoluto che ha caratterizzato i due anni che hanno preceduto questa legislatura, nei quali ben potevate avviare queste riforme, e non lo avete assolutamente fatto. Già è stato tratteggiato come si andrà articolando quella che non è una mini riforma ma qualcosa di molto di più. Intanto, per la prima volta, si è affrontato con determinazione e con lucidità uno dei grandi problemi del processo civile italiano: la molteplicità dei riti, ben 32. Entro 24 mesi si ridurranno a tre soltanto, di cui uno di nuova introduzione, il processo sommario di cognizione, un fattore certamente acceleratorio del processo. Abbiamo individuato una serie precisa di norme aventi un effetto deflattivo che favoriscono l'istituto della conciliazione con tutte le ulteriori conseguenze già ricordate e che per brevità non ripeto. Abbiamo dato per la prima volta tempi certi all'utente del servizio giustizia civile, infinitamente sfiduciato dall'interminabile lunghezza dei tempi, introducendo il calendario del processo. Abbiamo evitato - ed è stato giusto ricordarlo in questa sede - che decine, centinaia di migliaia di nostri artigiani e imprenditori perdano intere giornate di lavoro bivaccando nelle aule di giustizia per confermare soltanto una fattura, un documento di spesa non contabile. Abbiamo aumentato significativamente la competenza del giudice di pace, recuperando ulteriori risorse umane nell'autorità giudiziaria ordinaria al processo vero e proprio. E abbiamo introdotto il filtro che la Camera,

in sintonia con quanto avviene nelle altre grandi Nazioni europee, farà sì che l'unico giudice di legittimità italiano possa non essere soffocato da problemi infiniti, da questioni bagattellari, ma possa dedicarsi ai problemi più importanti. Onorevoli colleghi, questa per noi è la cultura del fare, la cultura di chi i problemi li affronta e li risolve e non continua eternamente a gestirli soltanto per farne materia di propaganda elettorale

Questa è la nostra cultura, la cultura del fare che è in sé un valore. Questa è la cultura che cambierà l'Italia.

il cui capo, *primus inter pares*, si intende ricevere con tutti gli onori in questo Senato. Spero che nel ricevere Gheddafi, però, non gli si dia il benvenuto a nome di tutti i senatori, come già è successo altre volte, perché ce ne sono molti che già si sono espressi contro la recente ratifica del Trattato tra Italia e Libia e altrettanti che hanno manifestato, anche attraverso dichiarazioni alla stampa, la propria contrarietà a continuare ad onorare questo signore.